Signor Presidente, vorrei brevemente aggiungere alcune considerazioni a quelle contenute nel testo della relazione. Il disegno di legge intende costruire le condizioni migliori per festeggiare degnamente il centocinquantesimo anniversario dalla morte di Gioachino Rossini, avvenuta a Parigi il 13 novembre 1868. Non credo sia necessario dilungarmi sulle ragioni che stanno dietro questa vasta volontà, tant'è universalmente noto a tutto il mondo Gioachino Rossini, così come il contributo da lui dato alla musica e alla cultura del nostro Paese e del mondo intero. Mi limito a dire poche cose, rimandando per gli aspetti più organizzativi alla lettura della relazione collegata al disegno di legge. Gioachino Rossini è stato sicuramente una figura eccelsa della creatività culturale e artistica dell'Italia; uno dei massimi esponenti della nostra tradizione lirica, ancora oggi invidiata nel mondo, e fattore dell'attrattività italiana, insieme a tante altre componenti. Rossini è stato un musicista originale, imprevedibile, per certi aspetti inafferrabile; un *mix* di arguzia e profondità, di buonumore e di slanci eroici. Ha saputo interpretare come pochi un tempo e un Paese. Ha interpretato il primo Ottocento e i suoi mutamenti. Dopo l'era classicista, dopo l'epopea di Haydn, Mozart e Beethoven, c'era una domanda di nuove emozioni, di nuove sensibilità; una richiesta di rappresentare idee e personaggi diversi, nuovi, e Rossini lo ha fatto, Rossini lo ha fatto, facendo parte di un movimento che poi ha portato al pieno dispiegarsi del Romanticismo musicale in Germania e in tutta Europa. Ha poi interpretato le doti dell'Italia, degli italiani e del loro carattere: la fantasia, l'allegria, la capacità di satira, la voglia di cantare, e anche i buoni sentimenti, gli ideali, le passioni grandi su temi grandi.

Penso ai due vertici assoluti: «Stabat Mater» e «Petite messe solennelle»: opere della maturità e della vecchiaia. In conclusione, le celebrazioni saranno utili sicuramente a ripercorrere la straordinaria parabola creativa di Rossini, ma sperabilmente anche ad altro. Penso essenzialmente a un affiancamento, importante e positivo per l'attività del Rossini opera festival di Pesaro, a cui va il nostro plauso per essere diventato ormai uno degli appuntamenti culturali annuali più importanti del nostro Paese; per provare a recuperare e valorizzare i documenti, gli archivi, i luoghi rossiniani che rappresentano comunque lo spaccato di un periodo significativo nella vita del nostro e più in generale a stimolare una nuova attenzione per l'opera lirica italiana in tutte le sue forme: quella comica, semiseria, seria, eroica, tragica. Rossini le ha visitate e praticate tutte e per questo è uno dei grandi nel *pantheon* della musica e della cultura italiana e mondiale. Vorrei concludere con l'auspicio che, accanto alle celebrazioni rossiniane, quest'anno, insieme alle altre realizzazioni fatte nel campo della cultura, possiamo mettere nel carniere anche altre realizzazioni significative, tra le quali vorrei citare la riorganizzazione del mondo dei conservatori e della formazione musicale, tanto attesa oggi nel nostro Paese. *(Applausi

bellezza neoclassica, purezza del segno vocale, vitalismo ritmico, il suo noto crescendo. Amante della bellezza in ogni sua forma, come della buona tavola, il compositore pesarese è stato capace - come pochi altri - di mettere in musica l'italianità. Nel 2019 si celebrerà la figura di Leonardo da Vinci (cinquecento anni dalla morte). Leonardo è l'icona del genio del Rinascimento italiano, l'ingegno multiforme, il talento poliedrico, la curiosità che non conosce barriere: pittore, scultore, inventore, ingegnere, scenografo, anatomista. Leonardo è una figura unica e inarrivabile: l'incarnazione dell'eccellenza italiana in ogni campo e in ogni forma. Il 2020 sarà l'anno della ricorrenza dei cinquecento anni dalla morte di Raffaello, il giovane e talentuoso pittore di Urbino. Raffaello è il pennello marchigiano che ha affrescato le stanze vaticane, che col suo sguardo profondo sull'animo ha dipinto un uomo nuovo. Le sue figure così vive lasciano a bocca aperta i suoi contemporanei. La sua modernità sorprende noi ancora oggi. Nel 2021 cadranno i settecento anni dalla morte del sommo poeta, il padre della nostra letteratura,

ma anche moderno, perché è sempre viva, in ogni uomo e in ogni epoca, la ricerca del ruolo da occupare nella società e nella storia. Come pure attuali sono le rinnovate domande che ognuno di noi si pone di fronte al mistero che avvolge l'universo e pervade il nostro microcosmo particolare. La lingua di cui parliamo è l'eco delle sue parole. Questo per dire che è giustissimo celebrare e ricordare figure che hanno fatto grande il nostro Paese e hanno portato avanti la nostra cultura E, per ricordarle, vengono istituiti dei comitati nazionali composti da esponenti di spicco della cultura italiana e internazionale, tutte figure di comprovata competenza e conoscenza. Si prospetta una auspicabilissima sinergia tra soggetti pubblici e privati. Si lavorerà alla digitalizzazione e alla condivisione delle opere di questi eccellenti artisti. È stata annunciata anche l'erogazione di borse di studio per i giovani studiosi interessati a tali opere. Se provvedimenti di questo genere non possono che essere appoggiati, tuttavia viene spontaneo mettere in questione la visione generale che è alla base di siffatte scelte. L'erogazione dei finanziamenti, infatti, non rientra in una visione politica e culturale organica, sistematica e coerente. Esportavamo cultura di eccellenza in ogni campo, ma oggi veniamo considerati analfabeti funzionali. Ce lo dice l'OCSE, che ci mette al primo posto di questa brutta classifica in classifica in Europa. Il 47 per cento degli italiani ha una mera capacità di analisi elementare ha una mera capacità di analisi elementare e, quindi, sono analfabeti funzionali e strutturali con una comprensione approssimativa. Gli antropologi e i linguisti dicono che l'Italia è, appunto, al vertice di questa classifica. Ci troviamo al di sotto del livello minimo di comprensione nella lettura e nell'ascolto di un testo di media difficoltà. la funzione e la capacità di comprendere. Spesso, non ce ne rendiamo neanche conto. Quasi un italiano su cinque lo scorso anno non ha mai aperto un libro o un giornale, non è mai andato al cinema o al teatro; non è mai andato a un concerto e neanche allo stadio e a ballare. Allora cosa facciamo facciamo noi in tutto questo? Istituiamo un comitato e rievochiamo il passato. Il nostro patrimonio culturale è una risorsa immensa, dalla quale dobbiamo attingere a piene mani. È la nostra ricchezza, sicuramente. Ma sa cosa mi viene in mente, signor Presidente? Mi viene in mente il detto di Maria Antonietta: se il popolo ha fame e non c'è pane, dategli delle *brioche*. Mi viene, quindi, da chiedere: gli italiani sono incapaci di ricostruire, di cultura, di approfondire? La realtà sfugge? sfugge? E allora, invece di dare un segno strutturale, un impegno verso la scuola, rivedendo tutti i gradi, dalle elementari fino all'università, noi formiamo i comitati. Una

spesi. Ci si chiede se questo sia il modo di risollevare il Paese e se c'è un ritorno. La settimana scorsa, signor Presidente, abbiamo celebrato Publio Ovidio Nasone.

Presidente, il mondo della scuola arranca; la nostra società è sempre più incerta e meno identitaria; le competenze vengono meno e le *fake news* trionfano su tutto, insieme a studenti svogliati e impenitenti, cui una volta mettevamo le orecchie d'asino, mentre adesso

abbiamo scuole con carenze strutturali, giovani sempre più disorientati e una culturale che fa sempre più fatica a emergere a livello internazionale. Cosa

o, parlando di Nasone, qualcuno lo confondesse con Pinocchio. Può capitare anche questo. Quando si guarda il particolare, non si guarda la sostanza delle cose. Pertanto, vorrei che qualcuno

non uno svilente ritorno elettorale per pochi. Meno marchette, più studio. *(Applausi dei

attribuire attenzione e, quindi, stabilire per legge un'opportunità unica nel panorama delle delle attività promozionali della cultura italiana all'interno del Paese e all'estero. Non dobbiamo dimenticarci, infatti, che c'è una valenza anche di natura

maniera indubitabile, l'Italia abbia un primato e una primazia che l'occasione del centocinquantenario contribuirà a rafforzare e corroborare. Ritengo che

Sono previsti concerti, mostre, attività didattiche. Ritengo, signor Presidente, che le mostre debbano essere itineranti, nel senso che non debbano fermarsi ai luoghi di nascita e di esecuzione della musica

in tutte le piazze e i teatri d'Italia, affinché questo evento rappresenti veramente un fenomeno globale e corale, in cui sia rafforzata - come dicevo prima - l'identità italiana, che pure è importante, non soltanto come uno spirito di natura patriottica,

Presidente, ritengo che a questo anniversario dobbiamo dare la massima importanza il Parlamento a occuparsene. Il Parlamento deve sfatare la vulgata messa in circolazione da quella superficialità di giudizio che - ahimè - anche tramite i *social network*, alberga in larghi strati della popolazione e che spesso vede nei giovani i soggetti sia recettori che proponenti. C'è in buona sostanza un'ignoranza di fondo che viene veicolata in quei circuiti, che va alla fine va alla fine a omologare tutto ciò che di positivo e di eccellente l'Italia potrebbe offrire. Con questi sentimenti

uno dei grandissimi e sommi geni tra i compositori italiani, che ha spaziato - come ben ricordato dal relatore - tra generi diversi, ma anche di aprire un canale di diffusione di quello che rappresenta la musica nel nostro Paese.

a garanzia di trasparenza, attraverso gli adeguati strumenti di comunicazione, quindi in termini più generali e non solo con riferimento al sito *web*. PRESIDENTE. Senatrice Blundo,

dichiarazione di voto.

parlando dell'emendamento. Ora, io vorrei capire.

ci è parso meritevole e condivisibile, poiché con esso si propone un'azione ad ampio spettro per favorire la migliore conoscenza, in patria e all'estero, dell'opera e della figura del compositore pesarese.

e agli orientamenti dell'epoca post-rivoluzionaria, proponendo un originale rapporto di autonomia tra musica e testo, facendo della sua opera un esempio culturale, capace di innovare gli schemi musicali e introducendo personaggi prima sconosciuti alle opere buffe. L'introduzione dell'ironia e del sarcasmo nel rigido modello settecentesco gli assicurò all'epoca un successo trionfale che è nostro patrimonio e che abbiamo il dovere di tenere vivo, per non disperdere ulteriormente un patrimonio culturale che ci è stato affidato dal tempo. La nota stilistica innovativa ha infatti dato lustro al nostro Paese in tutto il mondo e Rossini - descritto dai biografi come ipocondriaco, umorale e collerico, sovente in preda a profonde crisi depressive, ma anche gioviale, amante della buona tavola e di altre bellezze - è ancora considerato emblema e sinonimo di italianità. Queste poche e modeste parole, che spendo con ammirazione per ricordare la figura del grande maestro, ci spingono a plaudire al provvedimento in oggetto, poiché esso prevede, per il biennio 2018-2019, una condivisibile collaborazione tra enti pubblici e privati per realizzare numerose attività formative, didattiche, editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo per promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e documentario a lui riferibile. A ciò si aggiunga che la previsione del recupero e sistematizzazione dell'imponente materiale storico, artistico, archivistico e culturale riguardante il Rossini, nonché l'impegno per un intervento finalizzato al restauro dei luoghi rossiniani, anche con finalità di promozione turistica, rappresentano un provvedimento efficace ed un modello da proporre anche in altri provvedimenti. Purtroppo devo notare che, per quanto apprezzabile sia il cuore del provvedimento, ancora risultano particolarmente modeste le risorse stanziate allo scopo: la cultura, checché se ne pensi, è la radice dell'albero della nostra società e ha bisogno di sostanze per potersi rafforzare ed alimentarsi. che del provvedimento ci offre lo spunto per una ulteriore notazione di plauso è la previsione di borse di studio per l'elaborazione di saggi sull'opera di Gioachino Rossini da erogare in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali, della cui vitalità culturale in questi anni mi sono personalmente occupato. Ciò è importante perché il cammino verso la società della conoscenza e il miglior impiego della conoscenza, anche in economia, passano necessariamente per la valorizzazione, la condivisione e la divulgazione delle opere dei nostri concittadini migliori, che peraltro sono le più rappresentate, conosciute, citate e riprese dalla storia e nel mondo. L'ultima notazione positiva la riservo alla previsione di forme di divulgazione dell'opera del drammaturgo, da realizzarsi mediante l'utilizzo di tecnologie digitali. ovvio che tali impostazioni guardino finalmente avanti, verso il futuro: l'attuale conoscenza ha assunto una varietà di forme talmente sofisticate e diffuse nella vita quotidiana, oltre ad aver raggiunto una velocità di circolazione che solo pochi decenni fa appariva inimmaginabile. Ciò ci fa ragionevolmente sperare che gli strumenti predisposti possano far giungere l'eco dell'opera del grande maestro negli angoli più lontani del mondo, per seguitare a dar lustro all'Italia. Per

che siamo quello che siamo perché c'è chi è arrivato prima di noi e ci ha lasciato quell'altissimo livello culturale che ci permette di vivere e di essere la Nazione che siamo. Dovremmo quindi essere un grande Paese. Signor Presidente,

stiamo parlando di un provvedimento da 700.000 euro in due anni su una spesa totale dello Stato di 800 miliardi di euro. Siamo

ed economico: abbiamo problemi per quanto riguarda l'immigrazione e abbiamo problemi per quanto riguarda i nostri giovani che se ne vanno all'estero perché non trovano lavoro. Siamo in un momento in cui l'Italia è sotto gli occhi di tutti. Se andassimo a vedere

tutta l'Assemblea si stia predisponendo per celebrare degnamente questo grande italiano che tuttora dona all'Italia

tali ragioni, Presidente, il nostro voto favorevole è anche subordinato alla necessità che il Governo si impegni affinché tutte le iniziative predisposte, anche grazie al contributo straordinario di 680.000 euro più 20.000 nel 2019, possano dispiegare i loro effetti positivi su tutto il territorio nazionale. Le mostre devono essere itineranti,

all'estero, anche attraverso il coinvolgimento degli istituti di cultura italiana presso i nostri consolati e ambasciate, affinché la risonanza internazionale si tramuti in effetti

eclettico; florida la sua composizione, che ha spaziato un po' ovunque, dalle opere, alle musiche sacre. È un uomo moderno, riconosciuto precursore dei tempi, che ha associato capacità e versatilità. Era anche un uomo di mondo e non solo per le numerose mogli che ha

1-Movimento Democratico e Progressista esprimo il nostro consenso all'atto del Senato che dispone le celebrazioni dei centocinquant'anni dalla morte di Gioachino Rossini cui preme valorizzare l'opera del grande compositore italiano di origine pesarese. Ci sembra di particolare utilità il sostegno ad attività didattiche, editoriali e scientifiche legate all'Accademia rossiniana-Rossini opera festival e alla Fondazione Rossini, ma anche il recupero, il restauro e il riordino del materiale storico, archivistico, artistico e museale, insieme con il recupero edilizio e il restauro

Signor Presidente, egregi colleghi, la figura e l'opera di Gioachino Rossini hanno segnato profondamente la cultura e la storia del XIX secolo. A fronte delle innovazioni e dei valori di cui Gioachino Rossini si è fatto portatore, il testo all'esame di quest'Assemblea intende cogliere l'occasione dei centocinquanta anni dalla morte del maestro, che cade il 13 novembre 2018, per celebrarne la figura e le opere. Il disegno di legge originario ha subito una riscrittura importante durante l'*iter* legislativo, con la collaborazione dell'intera Commissione, cui va l'apprezzamento per lo spirito collaborativo e per l'unanimità dei consensi con cui ha licenziato questo provvedimento. Durante i lavori sono state, dunque, semplificate le procedure, rese più trasparenti le modalità di costituzione dei comitati promotore e scientifico e riallineate le risorse rispetto ad altri disegni di legge che, analogamente, prevedono celebrazioni di altre ricorrenze, come quelli relativi alla figura di Ovidio nonché di Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e Dante Alighieri. Nonostante la profonda riscrittura subita, l'obiettivo dell'articolato è rimasto pressoché immutato in quanto si propone di favorire la massima diffusione internazionale dell'opera e delle conoscenze legate a Gioachino Rossini e alla sua fortuna, attraverso progetti che presentino ampi e qualificati livelli di collaborazione fra istituzioni, istituzioni e scuole ed istituzioni e privati, sul piano nazionale e internazionale, valorizzando anche singole e autonome proposte a livello locale o di singole città. Le finalità degli interventi da realizzare nei prossimi due anni mirano al sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività formative (anche di carattere didattico), editoriali, espositive, congressuali, seminariali, scientifiche,

la conoscenza, anche mediante l'utilizzazione di tecnologie digitali, del patrimonio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Gioachino Rossini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale ed internazionale;

ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino, anche con finalità di promozione turistica. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario 4; *c)* promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi sull'opera di Gioachino Rossini, in favore degli studenti dei conservatori e delle accademie musicali; Per dare seguito alle finalità appena accennate viene istituito un comitato promotore. All'interno dello stesso è costituito un comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama ed esperti della vita e delle opere del compositore, con il compito di formulare le linee di indirizzo per le iniziative suesposte. Il contributo straordinario stanziato per l'organizzazione delle attività celebrative è quantificato in 700.000 euro per il biennio 2018-2019. Rossini non appartiene solo al nostro Paese ma al mondo intero. È importante che venga conosciuto ancora meglio: la celebrazione dei centocinquant'anni dalla morte sarà una grande occasione per diffondere cultura e ci sarà una struttura solida alle spalle su cui poggeranno tutte le iniziative. Rossini è l'ambasciatore di Pesaro e dell'Italia nel mondo. Pertanto, la sfida sarà coniugare l'alta qualità alla massima diffusione delle attività toccando le varie città rossiniane: oltre a Pesaro, anche Lugo di Romagna, Napoli, Venezia e Bologna, fino a Vienna e Parigi. Rossini verrà raccontato attraverso l'opera e la musica, il cinema e qualche contaminazione con il contemporaneo. È in occasioni come queste che la musica, il territorio e le persone si uniscono e l'Italia è capace di raccontarsi: il voto del Gruppo Alternativa Popolare sarà convintamente a favore del provvedimento. Signor Presidente, noi senatori di Sinistra Italiana riteniamo che sia giusto onorare la memoria di Gioachino Rossini nelle Aule parlamentari. Fare un gioco di priorità fra gli interventi, come ha fatto il senatore Centinaio, è un po' pericoloso. si indulge in questo ragionamento e lo si porta alle estreme conseguenze, si può finire in una situazione in cui i provvedimenti riguardanti la cultura e aspetti quali la memoria dei personaggi illustri sono relegati a ruoli sempre più marginali. Noi, invece, pensiamo che con la cultura si mangi e che con la cultura i territori del nostro Paese possano ripartire e che, anzi, Quindi, sostanzialmente, non devono mancare discussioni approfondite su questo argomento come non deve mancare il nostro sostegno a questa iniziativa. Poi, naturalmente, potremo discutere se questo obiettivo lo si realizzi bene o male ma, comunque, queste discussioni devono essere sempre ben presenti nelle Aule del Parlamento, in Commissione e in questa Aula.

una frazione non piccolissima e non trascurabile. Noi abbiamo voluto, per questo motivo, dare un segnale, come senatori di Sinistra Italiana, e, in occasione della votazione degli emendamenti, ci siamo astenuti sull'articolo riguardante la copertura,

si vuole celebrare poeti, musicisti e filosofi con dei disegni di legge che stabiliscono microfinanziamenti, per darne un finto lustro, in una mediocre guerra delle reliquie che si tramuta, nella reale quotidianità, in un'assenza di progetto e di visione d'insieme poiché manca una strategia lungimirante che sviluppi un impegno di ampio respiro nazionale. Senza un progetto culturale, che sviluppi interesse e ricerca, gli eventi sulla memoria, così come le targhe, risultano inutili. È come creare creare un parco giochi per bimbi senza giochi e, soprattutto, senza parco. Sì, perché i nostri parchi e le scuole rimangono ancora luoghi dove i poeti, i musicisti gli autori che hanno dato lustro alla nostra cultura sono relegati in polverosi stanzoni, nel migliore dei casi.

teatri disabitati, orchestre stabili divenute precarie, cinema chiusi, festival soppressi, zone archeologiche trascurate, monumenti e aree culturali che versano in un generale e vero e vero degrado non fa altro che convincerci che disegni di legge come quello in esame non servono. Queste celebrazioni dovrebbero essere un'occasione per ridefinire sicuramente delle priorità, tracciare una linea e delle prospettive di sviluppo, capire cosa sia davvero essenziale e cosa no, progettare

che non lasciano alcun segno, se non - appunto - delle reliquie ombrose. Il Movimento 5 Stelle ha preparato un programma di Governo dove cultura e istruzione sono i pilastri della società del futuro, in cui immaginiamo i cittadini liberi di conoscere e comprendere. Sul disegno di legge in esame il Movimento 5 Stelle si asterrà.

che tende a ricordare uno dei grandi italiani che ha dato un ampio contributo alla lirica italiana e a promuovere la cultura del nostro Paese in tutto il mondo.

della nostra Costituzione in materia di diritti dei cittadini e altre questioni? Pongo questo interrogativo perché credo che dovremmo sforzarci di individuare una modalità. Personalmente ritengo che il Governo possa far da tramite nel rappresentare la volontà del Paese nel ricordare questi grandi personaggi, magari riducendo il contenuto delle deleghe al Governo su questioni più importanti

Cosa dovrei dire su questo disegno di legge? Che un anno nazionale non si nega a nessuno, visto che nel 2018 celebreremo l'anno europeo del patrimonio culturale, di cui nessuno parla e per il quale sono previsti fondi cospicui da parte della Commissione europea. Ebbene, io non ho ancora visto uno straccio di programma da parte del Ministero

delle strategie messe in campo dal Ministero dei beni culturali per questa ricorrenza. Nel 2018, inoltre, il ministro Franceschini ha annunciato, dopo l'anno nazionale dei cammini e dopo l'anno nazionale dei borghi, l'anno nazionale del cibo: bene, un altro anno nazionale che verrà celebrato nel 2018. Oggi, con questo provvedimento, il Ministero dei beni e delle è ben ricordarlo, tutto è in mano al ministro Franceschini, che nominerà i componenti del comitato promotore, che a sua volta nominerà i componenti del comitato scientifico; *nulla quaestio* su questo, lo abbiamo fatto anche noi quando eravamo al Governo

spero l'Italia utilizzi, perché ha un patrimonio culturale vastissimo. Ma io non so nulla; forse voi sapete qualcosa, forse il presidente Marcucci ne sa più di me, ma personalmente non so assolutamente nulla.

decide i criteri? Li decide, naturalmente con un decreto, il Ministero, senza passare in Commissione. Va bene, lo abbiamo fatto anche noi, ma non vorrei che questi 700.000 euro - che non sono bruscolini - venissero dati al Rossini opera festival, alla Fondazione Rossini e all'Accademia rossiniana, che già prendono soldi dallo Stato, dal FUS, il famoso fondo unico per lo spettacolo. Cerchiamo di utilizzare questi 700.000 euro per

debiti pregressi, pasticci gestionali che appartengono al passato, ma per fare cose concrete con le scuole e con le accademie. Un'ultima osservazione.

il patrimonio culturale di questo immenso compositore e che i risultati siano certificati, visibili, tangibili; che i giovani possano avvicinarsi a questo personaggio straordinario, la cui musica è molto popolare e armonica, sentita vicina

Presidente, onorevoli colleghi,

anni dalla scomparsa di Gioachino Rossini sono un'occasione nazionale unica e rappresentano per la Regione Marche, così drammaticamente segnata dal sisma, anche un motivo di rilancio turistico e artistico. Per la mia città, Pesaro, che a Rossini ha dato i natali il 29 febbraio 1792, è il coronamento di un antico cammino che ha nella musica un radicamento profondo. L'importanza della ricorrenza rendeva necessario un apposito intervento legislativo per poter garantire una cornice adeguata ai tanti progetti e alle tante iniziative che verranno realizzate per ricordare una figura che seppe rinnovare il teatro musicale italiano e contribuì largamente a rinnovare anche quello europeo, segnando il futuro dell'opera e di tutta la cultura musicale. Le sue composizioni come «Il barbiere di Siviglia», «La gazza ladra», «La Cenerentola», «Semiramide» ed il «Guglielmo Tell» - solo per limitare le citazioni - sono patrimonio collettivo ancora oggi, e lo saranno domani, immortali e sempre attualissime, nella loro bellezza eternamente duratura. Quello stile dinamico, irresistibile nel tono caldo e passionale, a tratti irriverente e beffardo, capace di diventare satira di costume, che caratterizza la prima fase della produzione, riuscì ad aprire le porte del teatro anche alle fasce più popolari, prima di virare al sacro, quasi un ripiegamento dell'anima dell'artista nell'intimità dello spirito, con lo «Stabat Mater», composto fra il 1832 e il 1839, nella campagna parigina di Passy, dove il Cigno visse un lungo isolamento, ma anche una fase altamente feconda, scrivendo innumerevoli sonate, composizioni per piano, brani di musica da camera, prima della sua morte, avvenuta il 13 novembre 1868 a Parigi. Personalità complessa, genio assoluto della musica, Rossini rappresenta il volto dell'Italia nel mondo. Apprezzato, stimato e invidiato. Una carriera intensa, una grande produzione musicale, sempre segnata da una carica innovativa con la quale gli artisti a lui contemporanei sono stati obbligati a confrontarsi e anche a scontrarsi. Dall'opera buffa al melodramma, Rossini seppe dedicarsi in eguale misura ad entrambi i generi, rielaborando lo stile del Settecento e segnando l'Ottocento, riuscendo a fecondare con la sua capacità innovativa anche il tempo successivo. Decine di opere liriche musicate senza confini di genere, perché seppe appunto spaziare dalla farsa alla commedia, dalla tragedia all'opera seria e semiseria. Per questo abbiamo, di fronte a tale ricorrenza, un dovere quasi morale: celebrarla al meglio, riconoscendo al nostro Paese quella grandezza artistico culturale di cui, spesso, forse non siamo consapevoli nemmeno noi fino in fondo. Celebrare Rossini, per celebrarci, per dare valore alla nostra comunità al maestro così legata. Il 2018, come stabilito dal disegno di legge oggi all'attenzione di questa Assemblea, viene indicato come l'anno rossiniano e vedrà lo snodarsi dei tanti appuntamenti previsti fino al 2019. Esposizioni, seminari, lezioni, spettacoli - tutti dedicati al Cigno di Pesaro - potranno caratterizzare, grazie alla collaborazione di enti pubblici e privati, la vita culturale del nostro Paese, della Regione Marche, della città di Pesaro. L'Accademia L'Accademia rossiniana del Rossini opera festival insieme alla Fondazione Rossini daranno il loro contributo prezioso, come da anni del resto fanno, per poter promuovere in Italia e nel mondo la grande arte rossiniana. Accanto agli eventi, sarà possibile realizzare il recupero, il restauro e il riordino di tutto il materiale storico, artistico, archivistico e museografico riguardante la figura di Rossini, ma anche dei luoghi che, nella provincia di Pesaro e Urbino, gli furono cari, soprattutto il conservatorio. Nel suo testamento Gioachino Rossini nominò il Comune di Pesaro quale erede della sua proprietà, con lo scopo proprio di fondare e dotare quella città di un liceo musicale. Un ruolo centrale, così come ci insegna l'idea di una cultura intesa come motore della formazione proprio delle giovani generazioni, lo avranno gli studenti delle accademie e dei conservatori. Al comitato che il presente disegno di legge istituisce - presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri spetterà il compito di individuare le dieci figure che siederanno nel comitato scientifico. Sarà scritta - ne sono sicura - una bellissima pagina culturale di cui il Paese potrà essere orgoglioso. Infine, permettetemi di esprimere un sentito e doveroso ringraziamento agli autorevoli componenti del comitato promotore delle celebrazioni rossiniane: il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano; il dottor Gianni Letta, il presidente della RAI Monica Maggioni; un sentito ringraziamento va anche al collega, presidente della Commissione cultura, Andrea Marcucci e al relatore, collega Claudio Martini. Un ringraziamento giunge ovviamente in questa Assemblea anche dal Presidente della Regione Marche e dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Ringrazio, inoltre, ma non per ultimo, il ministro della cultura Dario Franceschini, in particolare per il sostegno dato a questo disegno di legge che rientra nel profondo investimento e nella grande attenzione riposte verso il mondo dell'arte, della musica, della cultura da questo Governo.

che è vero che esiste una legge, la n. 420 del 1997, che regola i comitati celebrativi nazionali e le edizioni nazionali,

- vi è la necessità espressa all'interno di questa norma, di lavorare in modo più ampio sul territorio nazionale e non con una programmazione che possa nel contempo coordinare queste tre grandi eventi, che avvengono nel 2019 per quanto riguarda Leonardo, nel 2020 per quanto

È vero che il comitato nazionale esiste e che quel capitolo non ha una sufficiente capienza, ma il lavoro di questi tre comitati che vengono istituiti, utili alla complessità della progettualità diffusa sul territorio nazionale e non, ci impone di fare un ragionamento specifico per questa operazione. Questi tre comitati collaboreranno tra loro e con il comitato storico-scientifico previsto dalla legge n. 420 per gli anniversari di interesse nazionale, al fine di divulgare e valorizzare un patrimonio culturale unico ed universale, superando possibili frammentazioni: quindi c'è anche un'ottimizzazione del lavoro. Lavoreranno alla realizzazione di un percorso mirato alla creazione di un'offerta culturale ricca ed eterogenea in termini di formazione, ricerca, divulgazione, conoscibilità delle opere di artisti, valorizzazione turistica dei luoghi ad essi legati e sviluppo delle competenze degli studenti nel settore dei beni culturali. Si istituisce a questo scopo anche una cabina di regia che è composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero I finanziamenti previsti, che sono in tutto 3,45 milioni di euro, di cui 450.000 euro che insistono sul bilancio dello Stato di quest'anno ed un milione per il 2018, 2019 e 2020 (quindi spalmati in quattro anni) saranno destinati alla realizzazione di progetti di ricerca scientifica, pubblicazione di materiali inediti, organizzazione di convegni, seminari, mostre e rappresentazioni teatrali, pubbliche letture ed eventi da svolgere nelle principali città e nei luoghi di vita e delle opere dei tre grandi artisti ricordati, con la massima attenzione, come dicevamo, al coordinamento con le università, con gli istituti e con le scuole di ogni ordine e grado.

C'è un punto particolare sul quale mi vorrei soffermare (poi naturalmente possiamo fare riferimento alla relazione, cui tutti i colleghi avranno sicuramente già attinto le loro informazioni). Mi riferisco all'articolo 6, che è stato introdotto durante

Stato-Regioni all'interno del comitati, che giustamente è stato accolto anche dal Governo, mentre l'altro è costituito dall'articolo 6, con cui si è inteso semplificare e razionalizzare le procedure volte a dichiarare un bene monumento nazionale che comunque nel tempo, anche recente, non si sono ridotte. Si veda ad esempio il riconoscimento come monumenti nazionali della Basilica palladiana nel 2014 e della Casa museo di Gramsci a Ghilarza (diversi decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministero dei beni e l'utilizzo di strumenti di vario rango normativo. Quello che si è verificato negli ultimi anni è che, in assenza di una specifica normativa (anche all'interno del codice dei beni culturali, che fa riferimento dichiarazioni di interesse culturale, ma non di monumento nazionale), si è evidenziata la necessità di una norma che andasse a dare una risposta a questa esigenza di carenza normativa. Quindi, al fine di superare l'eterogeneità delle soluzioni normative adottate, con l'articolo 6 si riconduce la dichiarazione di monumento nazionale a una delle tipologie di beni culturali previste dal codice, in particolare attraverso la modifica dell'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali, aggiungendo ad esso un periodo: «Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Cantini. Ne ha facoltà. Signor Presidente, non aggiungo niente rispetto a quanto detto dalla relatrice, se non alcune parole per quanto riguarda Leonardo. Leonardo di ser Piero da Vinci fu pittore, scultore, inventore, ingegnere, militare, scenografo, anatomista, pensatore, uomo di scienza; un personaggio dal talento universalmente riconosciuto, che più di ogni altro ha saputo incarnare l'epoca rinascimentale. Leonardo è l'icona del Rinascimento italiano, un genio a 360 gradi, che ci ha lasciato in eredità capolavori in tutti i campi in cui si è cimentato. Basti ricordare la Gioconda o le macchine volanti, per non dimenticare le scoperte scientifiche (come gli anelli di accrescimento delle piante) o gli studi anatomici sul corpo umano. Per la sua genialità, è difficile ancora oggi definire se sia un'artista o uno scienziato, ma è indubbiamente uno dei più grandi geni che l'umanità abbia potuto conoscere. Leonardo, oltre a rappresentare per antonomasia il genio, rappresenta anche nel mondo il Comune di Vinci e quella parte di territorio (l'Empolese Valdelsa, in provincia di Firenze) di cui Vinci fa parte, capace di custodire negli anni e soprattutto di valorizzare il patrimonio lasciatoci da questo grande personaggio. Un connubio così forte, quello tra Leonardo e Vinci, che è quasi impossibile non pronunciarli insieme. Nel corso degli anni questa parte importante della Provincia di Firenze ed il Comune sono stati capaci, attraverso un'offerta turistica integrata con il territorio, di preservare e valorizzare l'immenso patrimonio che Leonardo ci ha lasciato, offrendo a tutti noi la possibilità di apprezzarlo ancora oggi; un'offerta turistico-museale completa che, partendo dalla Casa natale di Leonardo, passando per il Museo leonardiano, dove attraverso un completo percorso espositivo si può compiere un vero e proprio viaggio alla scoperta della storia, della scienza e della tecnica e terminando poi con la Biblioteca leonardiana, ci dà l'opportunità di conoscere ed apprezzare il genio vinciano nella sua interezza. Questa nuova e completa offerta turistica è frutto di un lavoro fatto negli anni dalle amministrazioni locali, che ha permesso al territorio di conservare il patrimonio artistico, di aumentare le presenze turistiche e di generare un indotto economico importante per tutta l'area; un indotto economico sostenibile, in grado di creare nuove forme di occupazione, di formazione e di sviluppo. Chi ha visitato la Casa natale di Leonardo avrà potuto constatare quanto la bellezza e la grandezza delle opere e delle scoperte di Leonardo siano un tutt'uno con il paesaggio, con le dolci colline coltivate ad olivi di Vinci. Sono proprio questi esempi virtuosi che ci permettono di essere sempre più consapevoli delle opportunità offerte dal nostro patrimonio culturale dobbiamo essere altrettanto consapevoli che per valorizzarlo e renderlo fruibile oggi servono progettualità, competenze ed innovazione. Oggi, per promuovere e diffondere la cultura italiana non possiamo accontentarci di attrarre i turisti solo nelle città come Roma e Firenze o di affascinarli con opere di eccezionale bellezza come «L'ultima cena» di Leonardo da Vinci; occorre un'offerta culturale diffusa e interconnessa, capace di valorizzare la complessità del patrimonio artistico italiano. Per fare ciò è necessario che le amministrazioni locali a qualsiasi livello si convincano che il turismo può diventare un *asset* strategico di sviluppo socioeconomico, propulsore di ricchezza e di occupazione. Solo così potremo tornare a primeggiare tra le Nazioni capaci di attrarre, grazie alla ricchezza del proprio patrimonio, i grandi numeri del turismo culturale. Per questo penso che approvare oggi il provvedimento in discussione ci permetta innanzitutto di dare un giusto riconoscimento alle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, ma anche e non di meno di sostenere le amministrazioni locali impegnate da anni nella valorizzazione nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di questo grande italiano.

di contemperare la giusta celebrazione e il richiamo della comunità nazionale verso questi "mostri"

speriamo che ci sia oculatezza da parte dello Stato, e quindi del Governo che dovrà provvedere a inserire nel proprio bilancio

realizzeranno, sia a livello della comunità nazionale, che invece deve trarre il massimo vantaggio da queste celebrazioni. penso che sia altrettanto importante sottolineare la notevole valenza delle disposizioni contenute nell'articolo 6 di questo disegno di legge, ovvero quelle quelle inerenti la possibilità per le comunità e per gli enti locali e per le Regioni, di individuare e quindi indirizzare all'attenzione del Ministero una serie di eccellenze ed emergenze architettoniche, storiche e artistiche che rivestano le caratteristiche di monumento nazionale, cioè che siano emblematiche, paradigmatiche della cultura italiana e che possano fregiarsi di tale riconoscimento anche ai fini promozionali e della fruizione turistica. Questo mi sembra sia il contesto giusto per poter superare quelle enormi quelle enormi difficoltà che abbiamo avuto anche in 7a Commissione - che se n'è a più riprese occupata - quando giungevano, da parte di enti locali o di associazioni pubbliche e private, iniziative promozionali affinché un bene

la loro opera alla grandezza della Nazione. Pertanto è giusto che vengano riconosciuti come monumento e come patrimonio universale italiano, sia in Italia che nel mondo.

Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, alla ripresa dei lavori parlamentari, checché ne dicano i colleghi della Lega, è bene sottolineare l'importanza della calendarizzazione in Aula del provvedimento per le celebrazioni di Dante, Raffaello e Leonardo che, aggiungendosi alla riforma della disciplina dello spettacolo dal vivo e al disegno di legge per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Ovidio, dimostra la viva attenzione e la centralità data dal legislatore, da noi, ai temi della cultura. La costituzione dei comitati nazionali per celebrare coloro che rappresentano l'espressione della migliore cultura italiana, mira a costituire un percorso di valorizzazione a livello nazionale ed internazionale. È la tradizione culturale italiana che può trovare, con le disposizioni del presente provvedimento, un *input* propositivo di sostanza in occasione dei momenti celebrativi.

dei tre artisti attraverso l'integrazione e l'azione con il settore della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca. Ciò costituisce un fattore imprescindibile per raggiungere in modo adeguato gli obiettivi prefissati, ovvero la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di tre personaggi che sono emblema nel mondo del nostro patrimonio artistico, culturale e intellettivo. Ritengo, dal punto di vista logistico, che sarà fondamentale assicurare l'interazione e la collaborazione con gli enti territoriali e locali, sia in sede di elaborazione dei programmi generali di celebrazione, sia in quella di promozione delle attività da realizzare, in modo da poter offrire alle iniziative le giuste sinergie con i territori che storicamente e culturalmente sono legati alla vita e alle opere di Raffaello, Leonardo e Dante. La cabina di regia, istituita al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, avrà dunque un ruolo di coordinamento fondamentale tra i comitati istituiti a Roma, nell'ottica di un'offerta che non sia frammentata o scoordinata, e le realtà locali in cui, *in primis*, avranno luogo le espressioni celebrative, che peraltro sono una continuazione delle iniziative che si organizzano in queste città, a Ravenna in particolar modo, per ricordare i grandi personaggi che sono stati legati a questi territori. Uno degli obiettivi del provvedimento è promuovere iniziative di carattere internazionale che contribuiranno a una sempre maggiore e più profonda comprensione della nostra cultura, che, partendo dalle sue radici, ci riporta al nostro presente. L'occasione celebrativa, dunque, guarda all'estero, all'intero territorio italiano e alle sue articolazioni territoriali in un'ottica tripartita e unitaria insieme. È indispensabile dunque, anche ai fini dell'effettività di dare un'adeguata dimensione internazionale a tutti gli eventi, garantire il giusto spazio all'innovazione tecnologica per la divulgazione e l'esposizione di quanto si andrà a realizzare. In quest'ottica la tecnologia potrà metterci a disposizione un bagaglio di informazioni e notizie che trascendono le naturali In campo culturale, d'altra parte, è indispensabile esaltare la prospettiva di guardare oltre per valorizzare le doti artistiche, scientifiche o culturali dei nostri giovani, che, partendo dai temi proposti e dalle opere di Dante, Raffaello e Leonardo, possono trovare spunti di riflessione e di raffronto anche sulla nostra condizione attuale. Mi sia perciò concessa, infine, una breve digressione su Dante, le cui spoglie sono conservate nella mia città, Ravenna. A quasi sette secoli dalla scomparsa del sommo poeta fiorentino, avvenuta nel 1321, gli studenti italiani continuano a confrontarsi con le molte suggestioni offerte dalla «Divina Commedia», metafora del percorso personale che l'uomo, allora come oggi, si trova a compiere, e che, partendo dalla selva oscura del peccato, può condurre, attraverso la redenzione, alla salvezza. Parliamo del tema sempre attuale del viaggio che l'uomo compie, al confine tra bisogni e pulsioni personali, e le richieste che la comunità compie nei suoi confronti, che si traducono in convenzioni di convivenza, oggetto di ritrattazioni lungo il corso della nostra storia culturale. Non a caso, infatti, l'opera di Dante, con i temi da lui affrontati, che hanno appunto valore universale nel processo di identificazione delle persone, viene tradotta in quasi tutte le lingue del mondo. Appare dunque fondamentale che la ricorrenza del settecentesimo anniversario dalla morte del sommo poeta possa costituire un fertile terreno di dibattito e incontro, volto a ribadire l'imprescindibile ruolo svolto da Dante Alighieri, sia nella definizione della specificità letteraria italiana che nella costruzione di un immaginario che ha affascinato le culture di tutto il mondo. Far rivivere Dante nelle sue città, Firenze, Verona

nonché approfondire i temi e i contenuti di un messaggio poetico eterno, sulla scia dell'arrangiamento appena proposto, può permettere di trovare nuova risposta anche agli interrogativi che investono, in modo sempre più pressante, la nostra società. È questo che rende impellente l'incontro del nostro Paese e della nostra comunità con la figura di Dante Alighieri, con le sue opere e la sua viva creatività. L'incontro con Dante, d'altra parte, nel caso di Ravenna, rappresenta l'anima medesima della città. La città di Ravenna, benché abbia ospitato Dante solo negli ultimi anni della sua vita, davvero si identifica con questo poeta La rassegna di eventi «Ravenna per Dante», per fare qualche esempio, che raccoglie circa settanta appuntamenti nell'arco di tre mesi, attualmente in fase di svolgimento e prevede un susseguirsi di letture, traduzioni, incontri didattici, itinerari e cortei celebrativi, a dimostrazione della vitalità continua delle iniziative dantesche nella mia città, Ravenna. Anche il Congresso dantesco internazionale, inaugurato quest'anno, che si svolgerà con cadenza biennale fino al 2021, sintetizza la passione e la volontà delle istituzioni comunali nell'assegnare alla città ravennate un ruolo di primo piano negli studi danteschi. danteschi. L'obiettivo del disegno di legge, firmato da settantadue senatori provenienti da diversi Gruppi politici, che avevo presentato nel febbraio 2016 e che prevedeva un contributo straordinario per la promozione e lo svolgimento di iniziative in occasione del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri, pur partendo da una prospettiva decentrata, si prefiggeva in sostanza lo stesso obiettivo della proposta del Governo, ovvero potenziare quegli eventi celebrativi che sono uno strumento fondamentale per la conservazione e la divulgazione del patrimonio letterario dantesco di inestimabile valore. È questo lo spirito che anima le iniziative in corso a Ravenna e che dovrà coinvolgere il percorso che ci separa fino al 2021,

PLI))*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al nostro esame riguarda ancora tre illustri italiani, personaggi tra i più rilevanti della nostra storia e di quella mondiale.

Riteniamo importante che i tre distinti anniversari non siano lasciati all'azione isolata e purtroppo qualche volta frammentaria di distinti comitati per le celebrazioni, ma inseriti all'interno di un programma integrato e unico di iniziative storico-culturali che spettano proprio al nostro Paese,

ha anche la funzione di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della Nazione e sicuramente il ricordo e la promozione dell'opera di Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e Dante Alighieri rispondono pienamente al dettato costituzionale. Colleghi, risparmiamo l'apologia dei tre monumenti della nostra cultura. Potremmo discettare in questa sede per ore e giorni della loro opera, eppure non riusciremmo a rendere la loro grandezza. Essi, infatti, costituiscono

ulteriormente e far conoscere al meglio il valore di tale patrimonio nazionale. Grazie alle nostre decisioni odierne possiamo disporre che esponenti della cultura italiana e internazionale di comprovata competenza e conoscenza della figura da celebrare compongano i comitati citati in esordio. Sono peraltro previste benefiche sinergie tra rappresentanti di soggetti pubblici e soggetti privati che operano nel settore culturale e che abbiano maturato una speciale e comprovata competenza, nonché la conoscenza diretta della figura da celebrare. Nel dettaglio, il provvedimento prevede attività di restauro di oggetti o immobili sottoposti a tutela, nonché la promozione di attività di ricerca, editoriali, formative ed espositive. Sono previste anche forme di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica, per riuscire non tanto a dar lustro ai tre geni, quanto a far meglio conoscere precisamente, nel dettaglio, l'opera loro. In una prospettiva di internazionalizzazione, particolarmente felice ci appare la previsione dell'uso di strumenti digitali, come le piattaforme dinamiche *open data*, aggiornate e sviluppate attraverso le esplorazioni, per costituire i valori culturali da celebrarsi come patrimonio formativo, particolarmente in ambiti accademici e di ricerca internazionale, in modo che sia possibile utilizzare l'occasione celebrativa come forma condivisa di sviluppo educativo internazionale e come opportunità di esercizio di cittadinanza globale. La consapevolezza della divulgazione dell'opera di italiani eccezionali, i quali ben prima della Rete o del *web* hanno saputo farsi hanno saputo farsi precedere dalla propria fama al di là degli angusti confini nazionali, ci fa plaudire alla previsione, per i comitati nazionali, di un'azione da svolgere in stretto coordinamento tra di loro. A questo fine, ci pare misura di buon senso quella relativa all'integrazione e alla coerenza dei lavori dei singoli comitati con i programmi e le attività del comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le finalità saranno raggiunte mediante azioni condivise dalle diverse amministrazioni interessate, istituendo, per meglio riuscirvi, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, una cabina di regia formata da tre componenti, in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del MIUR e del MIBACT. Particolarmente importanti sono le disposizioni contenute all'articolo 6, che prevede la possibilità di dichiarare cose mobili o immobili come beni di interesse culturale, a chiunque appartenenti, se rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. In tal caso possono essere dichiarati monumento nazionale, così come lo possono essere quei beni che rivestano un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. Con questa previsione, per la prima volta, si sottopone anche il bene privato alle disposizioni di tutela dettate dal codice dei beni culturali, che viene novellato dal provvedimento. Il codice vigente, in ordine alla dichiarazione di monumento nazionale, non prevede una specifica procedura da porre in essere, limitandosi a stabilire che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale, «gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente» e, in altra parte, a far salve le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali. Purtroppo la novella proposta non riesce a chiarire tutti i dubbi in materia. Infatti rimane l'esigenza di chiarire se, e in quale misura, dalla dichiarazione di monumento nazionale scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla dichiarazione di interesse culturale. Si è quindi introdotta, forse con troppa fretta, una novella nel codice, prevedendo una procedura per dichiarare un monumento come nazionale, da includersi nella dichiarazione di interesse culturale, con la quale un determinato bene è riconosciuto come bene culturale. Non ci sfugge che il provvedimento in esame manca però di specificare se e in quale misura dalla dichiarazione di un immobile come monumento nazionale scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione sul medesimo immobile di interesse culturale. Si tratta di un aspetto non secondario, sul quale il Governo dovrebbe intervenire per il miglior coordinamento delle norme stesse ed eventualmente con un decreto attuativo *ad hoc*. Nonostante questa notazione, esortiamo il Governo ad agire, colleghi, l'iniziativa ci appare meritevole del sostegno del Gruppo Federazione della Libertà, che voterà a favore del provvedimento in discussione.

dedicare iniziative legislative alla cultura e agli italiani che hanno fatto grande l'Italia. Questo disegno di legge, che celebra i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio anni dalla morte di Dante Alighieri, anniversari che ricorrono, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021, prevede nel suo articolato la composizione di comitati,

nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono». Quello che mi auguro e che vivamente raccomando al Ministro

Vinci significa celebrare la culla del Rinascimento, una delle migliori espressioni della nostra Italia, che è arricchita ancora oggi del loro genio universale,

parole di riconoscenza e gratitudine da parte del nostro Gruppo. La celebrazione che però trattiamo in questo disegno di legge e che, confesso, mi sta più a cuore, è quella di Dante Alighieri. Come già ho avuto modo di dire nel mio intervento su Ovidio, con Dante Alighieri i nostri avi, come troppo spesso è accaduto, non sono stati lungimiranti.

italiana. Anch'egli, contrastato per la sua vita strettamente legata agli avvenimenti della politica, fu esiliato e non rivide mai più la sua patria. Quando si racconta la vita del poeta, raramente ci si ricorda che Dante ha vissuto per molti anni tra i monti dell'Appennino tosco-emiliano e tosco-romagnolo,

cosa per lui insolita. In quella antica famiglia marchionale trova ancora operanti i veri valori e comportamenti cortesi a lui molto cari.

Alighieri. Se qualcuno passa da quella terra, lo può andare a vedere perché è un'opera scultorea unica nel suo genere perché è il volto di Dante. Essendo vissuto in Lunigiana,

che al suo interno raccoglie sensibilità diverse, ma tutte convergenti nel riconoscere il dato celebrativo,

Mi preme anche richiamare l'attenzione dell'Assemblea su un aspetto che forse poco è stato messo in evidenza,

si articola. Mi riferisco chiaramente alla scuola, ai centri di progettazione e di esecuzione culturale quali le accademie, le università ed i conservatori, ai tanti centri studi, alla stessa società Dante Alighieri, agli istituti di cultura italiana all'estero, che potrebbero concorrere a creare una visione collettiva fondata

Queste sono le ragioni per cui riteniamo che il provvedimento abbia la dignità per essere discusso in un'Aula del Parlamento

Concludo facendo un rilievo che si riferisce al famoso articolo 6 della proposta di legge, ovvero alle disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale. Sembra quasi una foglia di fico; poiché sappiamo

con un provvedimento a parte, avremmo avuto l'opportunità di dare grande dignità a questa giusta esigenza da parte delle comunità locali, per veder riconosciuto un bene che appartiene alla propria storia e alla propria tradizione, elevato alla dignità di monumento nazionale.

ha finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché della valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico del nostro Paese. Questioni delle quali si discute forse troppo poco in queste Aule, per cui credo davvero che non sia stata assolutamente una perdita di tempo. In questo disegno di legge sono contenute disposizioni per le celebrazioni dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo e di Raffaello Sanzio e dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri. con il necessario anticipo, perché avverranno rispettivamente nel 2019, nel 2020 e nel 2021. Il provvedimento dunque offre i tempi adeguati per predisporre un programma celebrativo adeguato a dare risalto alla vita, al pensiero e alle opere di artisti considerati tra i più grandi geni dell'umanità. Peccato, come al solito, che alla congruità dei tempi non corrispondano adeguate risorse, che avrebbero dovuto essere aggiuntive e non andare a ridurre le già troppo scarse risorse assegnate al sistema museale, dando luogo, ahimè, a una semplice partita di giro, che ripropone il tema della scarsità delle risorse dedicate alla cultura nel nostro Paese. Ma trattandosi di un'occasione importante di valorizzazione della cultura e dei nostri territori, Articolo 1-Movimento democratico e progressista voterà a favore di questo provvedimento, anche perché i tre comitati previsti dal disegno di legge, forse un po' pletorici, essendo composti da ben quindici persone ciascuno, dovranno lavorare in stretta collaborazione nell'elaborazione del piano culturale e nella realizzazione delle conseguenti attività, in coerenza con i programmi e le attività del comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e con il coordinamento di una cabina di regia formata di regia formata da tre componenti, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, uno del MIUR e uno del MIBACT. A dire il vero, se non fosse che tutte queste persone coinvolte dovranno essere scelte fra esponenti della cultura italiana e internazionale

sinceramente mi sentirei di dubitare che un insieme di persone così numeroso possa davvero coordinarsi, lavorare insieme e dar vita a programmi che abbiano in comune attività di restauro, di ricerca, editoriali, formative, espositive e di innovazione tecnologica che possano divulgare in Italia e all'estero la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità di tre personaggi così importanti. Confidiamo dunque e vigileremo sulle capacità delle persone che saranno coinvolte e soprattutto confidiamo nella capacità di sintesi della cabina di regia e delle attività culturali e del turismo saprà effettuare. Sarebbe davvero un peccato sprecare un'occasione per creare lavoro per giovani studiosi e operatori del settore, per investire nella formazione sia scolastica che universitaria, per coinvolgere gli enti locali e valorizzare i territori in questione sono vissute e hanno sviluppato il proprio ingegno. Resta secondo me ancora da chiarire se, con la disposizione che dà al MIBACT la facoltà di integrare ciascun comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici o privati anche successivamente alla loro costituzione, si potrà andare oltre il numero dei quindici componenti e con quale periodicità i comitati devono inviare al Ministero i rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto. Quanto all'articolo 6, in materia di dichiarazione di monumento nazionale, anche secondo quanto segnalato dalla Commissione affari costituzionali, sarebbe stato opportuno chiarire se da tale dichiarazione scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla dichiarazione di interesse culturale prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Eppure, vite eccezionali come quelle di Dante, Raffaello e Leonardo meritano di essere ricordate e ripercorse anche andando oltre precisazioni e puntualizzazioni che ci porterebbero inevitabilmente a perdere tempo prezioso per il raggiungimento degli obiettivi che il

che sono da sempre la più efficace arma di pace, lo strumento più valido per il miglioramento della nostra vita e del nostro futuro. Ribadisco quindi il voto favorevole del Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista, con l'auspicio che i dubbi rimasti siano chiariti in corso d'opera e soprattutto che i soldi stanziati, anche se pochi, siano spesi in progetti seri, efficaci e trasparenti.

personalità che hanno raggiunto, nei loro campi di azione, risultati ineguagliati e che rappresentano, non soltanto per noi che siamo nati e viviamo nei luoghi in cui loro nacquero, vissero e operarono, ma per tutti i cittadini europei, un motivo di fierezza e orgoglio. Sono personalità dotate di risonanza internazionale e di notorietà, che hanno una capacità di suscitare ammirazione in tutto il mondo e che veramente hanno pochi eguali. Io credo che, di fronte a figure così straordinarie, sia stato corretto prevedere un'iniziativa legislativa non ordinaria, un disegno di legge caratterizzato innanzitutto dalla tempestività, quale si propone di programmare, fin da ora, iniziative che riguarderanno un triennio, dato che gli anniversari cadranno nel 2019, nel 2020 e nel 2021. di Alternativa Popolare voterà convintamente a favore, perché, come ha detto un grandissimo pensatore del Novecento, Von Balthasar: «In un mondo senza bellezza - anche se gli uomini non riescono a fare a meno di questa parola e l'hanno continuamente sulle labbra, equivocandone il senso

Noi dobbiamo, invece, valorizzare la bellezza, la nostra cultura e farla vedere a tutti, indicarla e sostenerla. È il patrimonio più grande che abbiamo, non ne abbiamo un altro così, e lo è da tutti i punti di vista, dai punti di vista umano, sociale e anche economico. Anche il nostro *made in Italy*, di cui ci riempiamo la bocca, nasce come frutto sul ramo della nostra tradizione culturale, artistica e musicale. Chi dice che con la cultura non si mangia sbaglia. È con l'ignoranza che non si mangia, e non certamente con la cultura. Oggi facciamo questa norma per ricordare tre monumenti del nostro grande patrimonio. La parola «monumento» ha la stessa radice di «memoria», ma la memoria non è un fatto del passato: è la vita e la forza del presente e del futuro. Per questo noi abbiamo il dovere di ricordare queste grandi personalità che hanno fatto grande la storia, una straordinaria storia, che è quella del nostro Paese. Il nostro grande patrimonio di bellezza è anche il più grande contributo che l'Italia possa dare all'Europa e al mondo intero, che non ne ha mai avuto bisogno come adesso, perché il mondo ha bisogno di bellezza, positività e di costruzione. Un altro merito che ha questo provvedimento - forse il primo e il più importante - mi sembra quello di avere messo l'accento sull'importanza di avere iniziative caratterizzate dalla sinergia.

nella quale trovino posto rappresentanti delle istituzioni, personalità eminenti della ricerca e tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo a fare proposte e a organizzare manifestazioni in un campo come questo. Mi sembra molto importante che con il disegno di legge al nostro esame si pongano le condizioni per una collaborazione proficua tra i comitati nazionali che si istituiranno e il comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, che opera dal 2013 presso la Presidenza del Consiglio. Credo, inoltre, che si debba sottolineare il fatto che, di fronte ad anniversari di questo rilievo, è importante che si organizzino manifestazioni in vari settori. Noi siamo chiamati a dare un impulso al settore scientifico, a quello della ricerca. Mi pare importante il richiamo alla necessità di valorizzare i luoghi in cui queste personalità hanno vissuto e operato. Mi pare importante il riferimento che si fa alla attività di alta formazione e all'attività di formazione scolastica. Mi pare importante il riferimento che si fa alle attività convegnistiche, seminariali, a quelle espositive, alla possibilità di utilizzare le risorse che sono state messe a disposizione per opere di restauro di beni mobili e immobili. Insomma, è un provvedimento completo, attento alla molteplicità di ricadute importanti che eventi celebrativi di questo tipo possono avere. Infine, osservo che nel provvedimento è anche adeguatamente rappresentata una necessità che ha ispirato l'azione del Governo e della maggioranza e che ha costituito una costante del lavoro che abbiamo svolto in ambito culturale in questi anni, e cioè la consapevolezza che ricordare in campo culturale ha senso se al ricordo si associa il guardare avanti; se, insieme alla esaltazione di un passato glorioso, si è capaci di indicare nuovi obiettivi, nuovi traguardi, nuove direzioni di studio e di ricerca, nuove conquiste da realizzare. me pare che nel provvedimento tale necessità abbia avuto una risposta adeguata e che questa consapevolezza sia pienamente presente. Noi abbiamo bisogno di una cultura che guardi non solo al passato, ma anche al presente e al futuro e sia una grande opportunità, soprattutto per i giovani.

con cui il Governo interviene molto pesantemente, colonizzandoli politicamente, sui comitati che dovranno occuparsi di realizzare gli eventi,

ben controllati, perché coordinati da una cabina di regia, di nomina diretta del Presidente del Consiglio, del MIUR e MIBACT, che sovraintenderà alle operazioni dei

Nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, così come nell'illustrazione che ha fatto la relatrice, il Governo e la stessa relatrice si affrettano a sottolineare come la legge n. 420 sia uno strumento inadeguato a finanziare il comitato per la celebrazione delle tre figure

ogni anno il Ministero riceve un certo numero di domande da parte di associazioni, movimenti o cittadini che vogliono costituire comitati per la celebrazione di centenari di personaggi illustri. Le domande, che vengono esaminate dal Ministro ogni anno, devono essere corredate da una relazione tecnica che deve recare gli obiettivi e il programma delle celebrazioni; l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie, distinte per fasi di attuazione; un bilancio preventivo delle entrate e delle uscite, redatto in forma analitica; un elenco di istituzioni, enti e studiosi coinvolti nel programma; una documentazione bibliografica aggiornata sui personaggi; proposte di designazione degli organi del comitato nazionale. Tutto questo deve essere presentato prima

Pensate inoltre che la legge n. 420 del 1997 può finanziare anche manifestazioni a carattere non esclusivamente locale; eventi o attività pluridisciplinari o plurisettoriali; può comprendere un piano economico che contenga voci di cofinanziamento da parte di altre amministrazioni o di privati; può finanziare reti di istituzioni culturali. Insomma, sembra proprio che questa legge abbia tutte le carte in regola per finanziare dei comitati, anche di grande spessore culturale come quelli di cui stiamo discutendo in questo momento. però competere. Bisogna presentare il programma prima e dire quello che si vuole fare prima. Bisogna competere con altre idee dello stesso tipo. queste idee vengono inviate al Ministero, che ha costituito la consulta permanente che giudica le proposte e che è formata da esperti del settore; una consulta a insediamento permanente che viene rinnovata ogni tre anni. A questo Governo però, signora Presidente, non piacciono le procedure per selezionare le idee migliori. Si preferisce intervenire per legge e posticipare il programma a dopo: prima istituiamo il comitato dei quarantacinque e poi vediamo quello che si deve fare, e loro decideranno dopo.

prevede la possibilità di non finanziare ulteriormente il comitato. E sì, c'è un giudizio: oh quale scandalo! C'è un giudizio sulle attività,

proprio in questi giorni stiamo discutendo del decreto di riparto dei fondi di questi miseri 463.000 euro, con la speranza di trovarne altri 700.000. Ad ogni modo, si tratta di un discorso che affronteremo in Commissione insieme ai colleghi e alla relatrice. legge è stata destrutturata. C'è un'idea ben precisa, c'è una regia dietro a tutto questo: basta con le procedure che selezionano le idee migliori; basta con gli orpelli; meglio fare leggi *ad hoc*, specialmente nella fase finale della legislatura. Meglio eliminare tutti i lacci e lacciuoli. Ecco dove stanno i tempi e le modalità non consone che ho letto nella relazione illustrativa del provvedimento. È questo il punto, signora Presidente: si sta destrutturando una legge sacrosanta che seleziona le idee migliori per provvedimenti *ad hoc* che spianano la strada sostanzialmente al Governo; spianano la strada della colonizzazione politica di questi eventi e soprattutto spianano la strada alle attività.

dove il ruolo dei privati non è precisato. Io sono favorevole alla partecipazione del privato nella elaborazione del progetto, ma qui sembra che ai privati chiediamo solo soldi. Anche sotto il profilo del contributo economico, però, non comprendiamo esattamente

abbastanza vicini nel tempo, nell'opera e nel prestigio. Quindi, avremmo anche potuto funzionalizzare il comitato rendendolo unitario. Ho visto, poi, che nell'articolato si prevede una collaborazione fra i tre comitati nazionali. Spero che vi siano una vera sinergia e - come scritto in mezzo ai commi in modo abbastanza distratto - anche una ricaduta per quanto riguarda il profilo turistico e culturale del territorio e del paesaggio. Sono, cioè, enunciati concetti importanti e, quindi, condivisibili, ma in un provvedimento scarno. Forse

una competizione fra i progetti. I progetti devono essere credibili e possono essere anche dedicati allo stesso tema. Può esservi il progetto A migliore del progetto B o il progetto C assolutamente inaccettabile rispetto al progetto B.

Ma se dichiarassi un voto contrario o finanche un voto di astensione, i giornalisti, che sono maliziosi, direbbero che Forza Italia è contro Dante Alighieri, contro Raffaello e contro Leonardo da Vinci. Quindi, dobbiamo far prevalere la *Realpolitik*. Per questo motivo, dichiaro il nostro voto favorevole nonostante tutti i rilievi che ho enunciato.

oggi ci accingiamo ad approvare una legge importante, volta a celebrare tre altissime figure della cultura italiana: Dante, Leonardo e Raffaello. Lo scopo di questa legge è quello di valorizzare in modo significativo a livello nazionale e internazionale, attraverso le attività di tre distinti comitati, il lascito culturale dei tre grandi, con iniziative di segno diverso, anche nei luoghi che videro sprigionarsi il loro genio, e con il coinvolgimento attivo dei principali studiosi a livello mondiale. Oggi, approvando in seconda lettura in quest'Aula questo provvedimento, noi sottolineiamo proprio un percorso che vede collaborare lo Stato con il mondo della cultura, con il mondo accademico e con gli enti locali, per sostenere di più e meglio la cultura. È un provvedimento, quindi, importante per noi tutti, per la nostra storia, per l'intero Paese in generale. È incomprensibile come alcune forze politiche siano state costruttive e abbiano votato a favore in Commissione e non lo facciano oggi in Aula. Avremmo auspicato un segnale diverso. Una riflessione, sì, che è stata sollecitata deve essere fatta. E dovremmo aprirla su come si possa rinforzare il percorso di valorizzazione senza dover procedere ogni volta

sarebbe buona cosa rifinanziare adeguatamente proprio per avere un luogo dedicato e sempre attivo che metta al riparo le celebrazioni dal rischio di un *iter* legislativo che, di volta in volta, potrebbe riservare improvvisi *stop*,

a riscoprirli e a trasmettere alle nuove generazioni la loro eredità culturale. Le eredità di Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e Dante Alighieri sono le fondamenta della nostra identità, che tanti fanno finta di difendere, ma che noi sosteniamo realmente anche con l'approvazione

colpisce molti lavoratori: la mancanza di sicurezza nei luoghi di lavoro.

in quel di Adria morivano presso un'azienda - la Co.Im.Po - quattro persone,

le difficoltà che molti lavoratori sono costretti a subire pur di riuscire a lavorare e portare a casa lo stipendio per mantenere la famiglia. ci fosse maggiore attenzione agli ambienti di lavoro. Mi rendo conto che ne parliamo spesso, ma nonostante tutto le cronache quotidiane ci riportano all'attenzione questo grosso problema,

129.000 lavoratori, 23.000 dei quali tra scienziati e ingegneri. In Abruzzo produce termocompressori per auto. di un'azienda attiva su numerosissimi settori: 80 diversificazioni, investimenti in 60 settori, immenso ritorno di utili. Per inciso informo che è attiva anche nella produzione di trizio per ordigni atomici, che dirige il National Security Campus (quindi testate atomiche statunitensi) e ha ricevuto finanziamenti per un miliardo e 271 milioni di euro da compagnie come Intesa Sanpaolo. In Italia ha spudoratamente sfruttato tutta la filiera di incentivi e ammortizzatori,

solo del profitto e a discapito degli interessi generali, ha sottomesso le istituzioni e la politica; la stessa politica che domani mattina, alle ore 9,30, andrà a sfilare e a promettere, come ha sempre fatto. I lavoratori sono in sciopero permanente dal 18 settembre e conoscono i politici, così come conoscono l'informazione nazionale che, ad oggi, è silente. Difendono le proprie famiglie, che pagano da ben nove anni il costante e ininterrotto utilizzo degli ammortizzatori, per una crisi del turbo che, di fatto, non c'è. Quella che c'è è, invece, una scelta ben precisa della *corporate*, atta a vanificare i continui sacrifici dei lavoratori. I volumi mondiali dei turbo Honeywell sono in crescita esponenziale. Altro che crisi! di scelte consapevoli, a discapito dell'Italia e a favore di Romania e Slovacchia, giustificate - si fa per dire - dal costo del lavoro. Solo tre anni fa vi fu un accordo modello - lo chiamarono così all'epoca - che regolò la gestione di 70 esuberi e pianificò un rilancio per l'anno successivo. Ad oggi è lapalissiano che l'azienda considera i lavoratori di Atessa come una semplice variabile all'interno di una logica in cui vi è solo il primato del profitto.

il piano per il polo di Atessa? Si ha forse paura di alcune conseguenze? Non è possibile che una multinazionale che fattura milioni di dollari e che continua a sfruttare la crisi, attingendo agli ammortizzatori da oltre nove anni,

Signora Presidente, desidero innanzitutto fare i complimenti alla magistratura e alle Forze dell'ordine per l'operazione condotta stamattina in Lombardia. La presenza della 'ndrangheta sul territorio lombardo e nella provincia di Monza e Brianza è nota da tempo, dall'indagine infinita del 2010. E io la denuncio da tempo. Su Seregno, in particolare, ho presentato nel 2015

Già in passato vi sono stati sequestri di droga e armi, oltre che chiusura di bar e altri esercizi commerciali per infiltrazione mafiosa. Alle mie interrogazioni il Governo non aveva ancora risposto; ora è urgente inviare la Commissione prefettizia di accesso e poi sciogliere il Comune per condizionamento mafioso.

perché è molto urgente che la 'ndrangheta trovi finalmente un baluardo nelle istituzioni, come è accaduto oggi. Mi associo quindi ai complimenti della collega alla magistratura e a tutte le Forze dell'ordine e insisto affinché il ministro Minniti destini più risorse per quella zona.

secondi sono pochi, ma sono interminabili quando svegliano una città nella notte; quando si vede tremare e crollare la casa e quando la gente si precipita fuori per paura di perdere la vita insieme ai beni e agli affetti più preziosi. Da allora, da quel 26 settembre, si sono susseguite varie scosse che sono durate mesi,

a gestire l'emergenza in modo encomiabile. Voglio poi ricordare Giancarlo Sagramola, ai tempi responsabile della Protezione civile nella mia città. E parlo della mia città perché è quella che